L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Onorevoli colleghi, si celebra oggi la Giornata della Memoria in ricordo dei milioni di vittime dell'Olocausto. Il Presidente del Senato si recherà oggi a Mauthausen a rendere l'omaggio della nostra Assemblea, deponendo una corona di fiori davanti al monumento alle vittime del nazismo.

restino solo come testimonianza e monito nei libri di storia.

Il primo richiamo che rivolgo al Presidente del Senato riguarda la necessità che le due massime cariche dello Stato, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, favoriscano un'intesa affinché l'attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il Copasir, non venga interrotta. in questa sede nel merito di polemiche politiche che sono in corso, che per primo non affronterò in Aula e che sconsiglio a tutti noi di affrontare, data la particolare natura di questo organismo, che ho avuto l'onore di di presiedere per circa due anni. Segnalo al Presidente del Senato, perché se ne faccia interprete, la necessità di considerare cosa stabilisce la legge a questo proposito. Questa mattina abbiamo dovuto prendere atto della inopportunità di svolgere una seduta già convocata per l'audizione del direttore del DIS

La legge stabilisce un criterio fondamentale, che è quello che il Comitato sia composto di un numero pari di membri di maggioranza e di opposizione e che la Presidenza sia affidata a un membro dell'opposizione, proprio per garantire il controllo il controllo su queste delicate attività. Stabilisce, inoltre, che la rappresentanza sia paritaria tra i due rami del Parlamento. In sostanza, vi devono essere cinque deputati e cinque senatori, così come - ripeto - prioritariamente ci devono essere cinque membri della maggioranza e cinque dell'opposizione in modo che, attraverso la parità, non venga consentito di determinare situazioni di maggioranze conflittuali su materie tanto delicate. Esiste poi un problema di rappresentatività, che ha conosciuto dall'inizio di questa legislatura molte mutazioni, com'è evidente e come accade in tutte le Commissioni bicamerali, poiché la instabilità politica nella composizione composizione dei Gruppi ha determinato e continua a determinare delle oscillazioni che, tuttavia, per prassi costante nella vita del Parlamento non sono tali da determinare violazione di quei due grandi criteri:

la nascita di nuovi Gruppi, l'equilibrio della composizione tra i Gruppi - che tuttavia non può portare ad una sostanziale soppressione dell'attività del Copasir. Ci rendiamo tutti conto che, prescindendo in

in rappresentanza dell'intero Parlamento di acquisire le informazioni che al Parlamento spetterebbero. La mia raccomandazione al Presidente del Senato è di lavorare nelle prossime ore assieme al Presidente della Camera per garantire che, anche laddove il problema serio della rappresentatività dei Gruppi non trovi una soluzione immediata, come già è avvenuto in altre fasi politico-parlamentari, non si arrivi all'impossibilità di svolgere le riunioni di un Comitato che è di importanza fondamentale per la vita delle istituzioni e per la capacità del Parlamento (poiché la legge stabilisce che sia quel Comitato a rappresentare ed acquisire elementi che non possono essere portati ad altre istanze con criterio di pubblicità), impedendo, quindi, che questa attività venga interrotta: questo non ce lo possiamo permettere. Il mio intervento, quindi, non è un richiamo alla polemica politica, né alle vicende che riguardino l'uno o l'altro Gruppo, tutte rispettabili, ma è una sollecitazione affinché il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, faccia in modo che questo Comitato, pur in attesa di una compiuta definizione dei criteri di rappresentanza, possa riunirsi, anziché dovere rinviare e cancellare le proprie sedute, in un momento di tale delicatezza politico-istituzionale.

faccio mia, a nome del Gruppo che rappresento, la preoccupazione espressa dal senatore Rutelli. Vorrei solo fare una precisazione, che tra le altre cose si evince dalle parole che il senatore Rutelli ha usato.

si stabilisca poi un criterio proporzionale per la rappresentanza dei Gruppi, all'interno della maggioranza e dell'opposizione. Ciò che assolutamente non può venir meno, altrimenti l'organismo si verrebbe a trovare in una situazione di illegalità, è il criterio di parità tra maggioranza e opposizione,

Il problema si è creato alcuni mesi fa, nel momento in cui sono cambiati i rapporti interni all'allora maggioranza, per la formazione di un altro Gruppo, che proporzionalmente non aveva diritto

parità tra maggioranza e opposizione, mentre il criterio di rappresentanza all'interno della maggioranza e dell'opposizione,

ci si deve rifare alla situazione originaria, non tenendo conto delle mutevolezze della legislatura. Questa è stata l'interpretazione che hanno dato insieme il presidente Fini e il presidente Schifani. Si è posto un ulteriore problema nel momento in cui una forza politica che faceva parte della maggioranza è passata all'opposizione. In quella circostanza, un componente di quella forza (il FLI), l'onorevole Briguglio, ha presentato, correttamente, le sue dimissioni, per consentire che la parità tra maggioranza e opposizione si ripristinasse. Cosa è accaduto? Tenendo conto della loro stessa dottrina, esposta - come ricorderà la collega Finocchiaro - in una Conferenza dei Capigruppo, i presidenti Fini e Schifani hanno scritto ai Gruppi, tenendo conto della situazione originaria e Il problema è sorto nel momento in cui il Gruppo al Senato a cui è stato scritto ha ha fatto la propria designazione, laddove la designazione del Gruppo alla Camera del PdL è stata bloccata. Dunque, in questo momento, senatore Rutelli, il Copasir viene a trovarsi così composto: cinque membri di opposizione più un dimissionario, quattro membri di maggioranza. Viene meno quel criterio di parità senza il quale un organismo così delicato viene a trovarsi in una situazione di illegalità. Questo, evidentemente, perché è mancato un raccordo all'interno dei Gruppi di opposizione: lo dico sommessamente, senza su questo voler sviluppare alcun tipo di polemica. Alla luce di queste considerazioni, che sono la pura verità, è evidente che l'organismo, per tornare a lavorare - ed è bene che lo faccia immediatamente deve ristabilire quella condizione che la legge fissa come assolutamente imprescindibile: parità tra maggioranza e opposizione. Ed è per questo che al suo invito, cioè all'invito presentato ai Presidenti di Camera e Senato per trovare degli accordi, aggiungerei anche, sommessamente, un invito ai Gruppi dell'opposizione affinché si possano verificare tra loro quelle intese che portino a ripristinare una parità. Faccio presente che, nel momento in cui queste intese nella maggioranza non erano state raggiunte, pur in presenza di criteri proporzionali chiaramente falsati, proprio in considerazione dell'importanza e della delicatezza del Copasir, il Gruppo del PdL disse apertamente che, pur non essendo d'accordo e volendo investire della questione la Giunta per il Regolamento, avrebbe comunque continuato a partecipare ai lavori dell'organismo, proprio per garantirne la vita e l'operatività. Io spero che lo stesso Io spero che lo stesso atteggiamento di responsabilità si possa riscontrare - lo dico senza polemica - tra i Gruppi dell'opposizione affinché si possa ripristinare quella condizione di legalità senza la quale,

per forma di cortesia istituzionale, non replico al presidente Quagliariello. Prendo atto della sua dichiarazione per cui il Presidente del Senato cercherà di farsi carico, così come ovviamente le opposizioni provvederanno, visto che la situazione è cambiata nelle ultime ventiquattrore tra Camera e Senato, a designazioni inequivocabili che consentano però - ripeto - la funzionalità dell'organismo. Chiedo, invece, di intervenire, signora Presidente, per rivolgere un richiamo alla Presidenza del Senato e al Governo, qui rappresentato dal Ministro degli affari esteri e da altri autorevoli membri, perché la seduta di oggi, a mio modo di vedere, si occupa di una materia che rischia di creare un precedente che non si è mai registrato nei rapporti tra i due rami del Parlamento.

il suo predecessore, mentre il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di un dibattito su una materia, di «straordinario» interesse politico, istituzionale ed economico, riguardante un'eredità confluita

competenti giurisdizionali, poiché è in corso un'indagine della magistratura che dovrà dare i suoi frutti, così come mi auguro avvenga su molte altre questioni che sono oggi oggetto della discussione politica pubblica.

del Presidente della Camera dei deputati? Bene, penso che sia la Camera che il Senato dovrebbero avere su questo il senso di responsabilità di non creare un precedente che in questi decenni non si era mai creato. Voi, oggi, con la decisione, assunta dal Presidente del Senato, di fare questa discussione obliqua sul Presidente della Camera, a pretesto di un'interrogazione del collega Compagna presentata in poche ore e in pochi minuti messa all'ordine del giorno del Senato, non affrontate un tema che noi vogliamo non affrontare, perché non abbiamo nessun problema: si affronti, si svisceri e si discuta tutto quello che si vuole, sulla materia della casa di Montecarlo e di non so quali altri aspetti riguardanti l'eredità della signora Colleoni. Ma non ci si venga a dire che questo sia un modo per affrontare, con la presenza del Ministro degli affari esteri,

un'esposizione riguardante la situazione politica nel Nordafrica. Certo, se si fosse presentato nell'Aula del Senato soltanto per parlare della rogatoria dell'autorevole Stato di - come su un'abitazione che si trova in Montecarlo, credo che il rappresentante della sesta potenza economica del mondo non avrebbe motivo per essere particolarmente orgoglioso, visto ciò che sta capitando a livello internazionale. Ha avuto, quindi, la decenza di allegare all'importante tema della casa di Montecarlo l'esame della gravissima situazione nel Nordafrica. Vorrei, signora Presidente, che il Senato della Repubblica fosse consapevole che ciò che avviene questa mattina non avrebbe dovuto avvenire, per la correttezza dei rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Io mi sono dimesso Io mi sono dimesso dalla Presidenza dell'organismo del quale parlavamo prima per un motivo di opportunità politica, ma questo non c'entra proprio nulla con la richiesta di dimissioni che viene rivolta al Presidente della Camera nell'altro ramo del Parlamento. Nel mio caso, aver mutato l'appartenenza politica avrebbe potuto assoggettare un organismo di quella delicatezza, che opera sotto regime di riservatezza e segretezza, a problematiche improprie. In questo caso stiamo parlando della terza carica della Repubblica, che ha una funzione non stiamo parlando quindi di qualcosa che non è mai avvenuto: è avvenuto tante volte nella storia repubblicana.

infedelmente, in modo irrispettoso della Costituzione e dei Regolamenti del Senato della Repubblica, e lo stesso può avvenire alla Camera dei deputati; ma che il Senato della Repubblica si occupi in maniera obliqua della polemica interna alla Camera dei deputati, prendendo a pretesto una materia per la quale, secondo me, se il Ministro degli affari esteri avesse avuto la dignità di mandare

è stato per senso di responsabilità di tutti i Presidenti che lo hanno preceduto, e se oggi lui accetta che si faccia per vie traverse un dibattito sul Presidente della Camera compie un errore. In conclusione, signora Presidente, vorrei

su cui prende ora la parola. Le comunico anche che, terminata questa discussione procedurale, per non prestarmi a questo dibattito che considero inaccettabile per i profili che ho delineato, non ascolterò l'intervento del Ministro degli affari esteri.

Il mio intervento è necessitato dall'urgenza, io credo, di evitare che uno scontro politico si trasferisca in una sede istituzionale, e che la sede istituzionale, i suoi Regolamenti, i suoi tempi e i diritti dei componenti l'Assemblea vengano piegati a contingenze di natura politica, particolari e estranee al dibattito in corso in questo ramo del Parlamento. È ovvio che questo richiamo al Regolamento implica decisioni e responsabilità diverse. Il mio Gruppo ha tentato di fare un esame del numero delle interrogazioni a risposta urgente giacenti

Dall'esame che i miei uffici stanno conducendo emerge che il *software* del Senato indica circa 1.800 interrogazioni giacenti: tra queste, è difficile sceverare, se non con un'analisi testo per testo, quali siano quelle a risposta urgente, ma certamente ci muoviamo nell'ordine dei grandi numeri. Sappiamo benissimo che esiste una valutazione da parte della Presidenza del Senato circa il carattere di urgenza dell'interrogazione che viene proposta, che è di natura discrezionale e, naturalmente, di natura squisitamente politica. L'urgenza si collega normalmente a fatti che interessano la collettività, che sono di rilevante interesse nazionale e rilevante interesse pubblico.

che l'interrogazione del collega Compagna, presentata il 25 gennaio, in orario successivo alla Conferenza dei Capigruppo, fosse tale da necessitare

Questo, mentre alcune grandi questioni che attengono alla vita del nostro Paese, ai destini del nostro Paese, alle condizioni materiali di vita di milioni di italiani e di italiane, che sono condensate in interrogazioni presentate, giacciono perché non se ne è ritenuta l'urgenza. Il collega Rutelli diceva che il ministro Frattini ha colorato questa sua presenza con

Innanzitutto, che la presenza del ministro Frattini qui è stata necessitata dal fatto che prima il mio Gruppo e poi altri hanno presentato delle interrogazioni esattamente sul tema che riguarda le vicende internazionali che coinvolgono la Tunisia, piuttosto che l'Egitto, l'Albania o l'Algeria (adesso si sono aggiunte altre due interrogazioni che focalizzeranno meglio i punti della discussione).

ad un'interrogazione la quale avrebbe, casomai, necessitato che a riferire qui in questa Aula, rispondendo all'interrogazione, fosse il Ministro della giustizia e non quello degli affari esteri. Perché faccio questo discorso e perché sto insistendo su questo punto? Certo, siamo assistiti dal parere espresso autorevolmente, esattamente in queste ore - potremmo dire - dal Presidente della Repubblica che invita tutte le forze a non trasferire gli scontri politici nelle sedi istituzionali. Però mi sento di aggiungere un'altra cosa, e cioè che a questo va connesso un altro tema: quello del diritto delle opposizioni di vedere discutere le loro interrogazioni in Parlamento. Questo è un punto essenziale. Non è possibile che, per piegare l'Aula del Senato, la discussione, la stessa presenza del Governo in quest'Aula ad un'esigenza di natura squisitamente politica e - lasciatemi dire - assolutamente insignificante rispetto ai problemi che ha il Paese in questo momento, il Ministro degli affari esteri venga convocato, questa interrogazione venga messa immediatamente all'ordine del giorno, mentre decine, centinaia, non so se migliaia di altri atti ispettivi che riguardano questioni assai serie che vengono proposte dalle opposizioni giacciono e, probabilmente, non avranno mai una sede, un'occasione, un interlocutore per discuterne e per manifestare anche la qualità del lavoro e della presenza sui temi della politica generale dei Gruppi di opposizione.

signori del Governo, credo che le riflessioni che hanno appena sviluppato il senatore Rutelli e la senatrice Finocchiaro rendano inutili alcuni riferimenti che pure avrei voluto fare, con richiami al Regolamento e all'ordine dei lavori.

l'ultima volta che un Ministro è stato qui per rispondere ad un'interrogazione, in quel caso a risposta immediata,

le istruttorie, e poi i processi, come deve essere, in particolare quando si tratta di soggetti pubblici che hanno un ruolo istituzionale importante. Non è in discussione l'esigenza di chiarezza e di trasparenza, se il dibattito parlamentare anche su questi temi non fosse inficiato dalla strumentalità e dalla subalternità delle istituzioni alle esigenze di lotta politica.

con qualche difficoltà da parte della maggioranza a mettere insieme il numero legale, perché questo avrebbe significato impedire il confronto parlamentare. Noi vogliamo invece che

una capacità di lavorare in tempo reale: sarebbe una straordinaria pagina parlamentare, se questo diventasse la regola. Vi immaginate? Una capacità di risposta del Governo in tempo reale, in ventiquattrore, sulle grandi questioni, sui grandi problemi e sui grande temi!

soggetti, mi interrogo con un po' di umiltà sul punto - se ed in che misura interagisce ed interferisce rispetto a questa calendarizzazione il ruolo del Presidente del Senato.

il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148». Cito

del Giorno della Memoria. Credo che nel silenzio, dentro di noi, tutti abbiamo sentito la colonna sonora de «La vita è bella»;

ricordato il collega Viespoli, siamo in presenza di un'interrogazione che su, richiesta dell'interrogante (così come recita l'articolo 151 del carattere d'urgenza. Tale richiesta viene riconosciuta come tale dal Governo, che si dichiara pronto a rispondere in tempo reale; la valutazione finale sull'urgenza di questo atto pseudo-ispettivo viene fatta insindacabilmente dal Presidente del Senato, il quale si è assunto la responsabilità di ammettere un'interrogazione

attraverso una procedura che non è quella prevista rispetto ad un procedimento penale in corso, che coinvolgerebbe l'utilizzo dello strumento della rogatoria internazionale, e quindi il ruolo del Ministro della giustizia;

In realtà, si tratta di un atto che, ancorché formalmente non citi il presidente Fini, riguarda un'indagine in corso, di cui tutti siamo rispettosissimi. Magari fossero tutti rispettosi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura come lo si è in questo caso, perché ciò darebbe veramente molta serenità a questo Paese. molta serenità a questo Paese. Siamo in presenza di un giudizio di ammissibilità che fa precedente e che viola il Regolamento, portando il Presidente del Senato a venir meno al suo ruolo di terzietà e di imparzialità rispetto all'andamento dei lavori

che devono restare terze, in una lotta politica che oggi è obiettivamente intollerabile, insopportabile ed indecente. Per tali ragioni, noi abbiamo detto che l'ammissione di questa interrogazione è un atto di indecenza dal punto di vista istituzionale, che viola l'articolo 151 del nostro Regolamento e apre, obiettivamente, la strada ad un conflitto istituzionale di cui nessuno di noi sente il bisogno. Mi permetto inoltre di aggiungere che anche anche dal punto di vista politico - lo dico senza polemica ai colleghi di maggioranza - è un atto scorretto nei confronti degli altri Gruppi parlamentari. Infatti, al di là delle questioni già poste, e da me condivise, dalla collega Finocchiaro e dal collega Viespoli, c'è un punto centrale della vicenda che dobbiamo avere sempre presente: l'utilizzo dell'articolo 151 del Regolamento, così come operato dalla maggioranza e dal Presidente del Senato, determina l'assenza di un contraddittorio rispetto alla questione politica e trasforma l'interrogazione a risposta orale urgente in un *question time* camuffato, senza la possibilità della partecipazione degli altri Gruppi parlamentari a questo dibattito,

se veramente volevate fare la forzatura, facendo venire in questa sede il Ministro degli affari esteri, dovevate utilizzare l'articolo 151-*bis*, anche perché *question time* in quest'Aula, purtroppo, non se ne fa da troppo tempo.

che abbiamo in più occasioni denunziato. Le prerogative dei parlamentari si esplicano essenzialmente in due modi;

abbiamo dovuto purtroppo lamentare in più occasioni che si è abbastanza radicata una consuetudine per cui

prevede che agli atti di sindacato ispettivo si risponda entro un termine di 15 giorni.

dell'articolo del Regolamento che prescrive un termine di 15 giorni. Abbiamo poi delle interrogazioni cosiddette assistite da determinate procedure. Nello stesso ordine del giorno di oggi vi è l'interpellanza

la corsia preferenziale prevista dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, ossia il procedimento abbreviato,

ha avuto il privilegio di una corsia privilegiata, con la procedura cosiddetta abbreviata, per cui, dal 18 novembre 2010, nell'arco di

non risulta peraltro come rientrante nella categoria delle interrogazioni urgenti.

vorremmo capire se la predisposizione dell'ordine del giorno è stata fatta per rispettare le prerogative del Senato e i diritti di ciascun senatore a porre questioni di sindacato ispettivo e ottenere risposte dal Governo o se obbedisce a un'altra logica. Ma siamo diventati una piazza o siamo sempre il Parlamento? Insomma, rispettare il Regolamento significa rispettare le regole, significa rispettare i parlamentari! Siamo stati violentati a termini di Regolamento, attendendo da anni risposta alle interrogazioni. E ora, solo perché fa comodo politicamente, un'interrogazione presentata l'altro ieri viene subito posta all'ordine del giorno!

non posso entrare su tutti gli aspetti del dibattito regolamentare che si è svolto. Mi permetterei, però, senza violare la la norma regolamentare che prevede che l'interrogante abbia la parola soltanto dopo l'interrogato, di fornire qualche precisazione,

Le ragioni che hanno mosso la mia interrogazione sono contenute nel testo, e non commetterò la scorrettezza parlamentare di servirmi di un richiamo regolamentare per illustrarle. Se si legge quel testo, e si ha memoria serena della documentazione giornalistica di quel giorno, di ieri, di oggi,

fattorino di *dossier* fabbricati, o millantati di fabbricazione, o diffusi con gli strumenti privatissimi del cosiddetto giornalismo investigativo.

che gli intenti della mia interrogazione e le ragioni per le quali, nell'ambito del mio Gruppo, ho creduto di avere il diritto, ma forse anche il dovere, di presentarla io sono diametralmente antitetici al processo alle intenzioni celebrato in questa discussione regolamentare. Per esperienza politica e personale non ho mai fatto parte del partito politico dal cui asse patrimoniale ha iniziato a svilupparsi una vicenda internazionale. infatti, ha assunto un profilo internazionale tra il Principato monegasco e l'isoletta di Santa Lucia non solo in questi ultimi giorni, ma quando, mesi addietro, si è parlato di privatissimo giornalismo investigativo organico al Governo teso a fabbricare dossier. comunque, non posso accettare, colleghi, che l'unico canale istituzionale di queste vicende debba essere quello della magistratura. Esiste un canale istituzionale

Voglio dire soltanto che il canale della magistratura lo rispetto talmente che uno degli avvocati dell'onorevole Gianfranco Fini, terza carica dello Stato, da me mai evocata nel testo dell'interrogazione, è una persona a me carissima: è mio figlio.

la invito a concludere. COMPAGNA *(PdL)*. Se il mio è stato un pasticcio, penso che il Regolamento me ne fornisse la possibilità. Se da parte di qualcuno c'è stato un eccesso di zelo nella calendarizzazione, avrei accolto con grande rispetto,

So però, per quanto riguarda la mia personale esperienza, che a suo tempo si è consumata la revoca e lo scioglimento della Commissione bicamerale di vigilanza, alla Presidenza della quale fui eletto democraticamente con voto segreto, e anche quella è una vicenda mai accaduta in precedenza.

le ragioni politiche su quelle giuridiche, valide e consistenti, come lo stesso presidente Fini autorevolmente mi ricordò. In definitiva, ascolto con rispetto

questo per far rilevare che evidentemente siamo in una legislatura per così dire costituente e che non ce ne siamo accorti.

cui risposta potremo avere immediatamente. Abbiamo appreso dai giornali che il Ministro degli affari esteri avrebbe trasmesso la documentazione proveniente da Santa Lucia alla procura della Repubblica di Roma. Così facendo, egli ha assegnato alla documentazione pervenuta al Ministero degli affari una particolare caratteristica disciplinata dalle norme della procedura penale.

una particolare condizione di segretezza che attiene ai documenti trasmessi all'autorità giudiziaria: da quel momento non se ne ha più la disponibilità. Vorrei sapere dal Ministro degli affari esteri se i documenti dei quali intende in questa sede parlare sono gli stessi trasmessi all'autorità giudiziaria e se si sia posto, quindi, il problema della violazione del segreto di indagine.

l'onorevole Giovanardi eccepiva le argomentazioni sviluppate dal collega Li Gotti in merito al fatto che sui giornali esista una diffusione del contenuto dell'atto. Questo varrebbe, immagino, a parere dell'onorevole Giovanardi, ad eliminare il vincolo del segreto istruttorio. Mi permetto di ricordare in quest'Aula che la diffusione di una notizia avvenuta illegittimamente non solo non elimina il vincolo del segreto, ma casomai rende responsabili in ordine alla diffusione di notizie coperte dal segreto. Credo che fosse esattamente questo il senso dell'intervento del senatore Li Gotti

ringrazio, senatrice Finocchiaro. Credo che il Ministro abbia ascoltato sia l'intervento del senatore Li Gotti che quello della senatrice Finocchiaro.

l'ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo secondo i criteri stabiliti nel Regolamento e alla luce della prassi parlamentare.

del senatore Morando)*. Pertanto, ritengo che un giudizio di inammissibilità da parte del Presidente del Senato sarebbe stato oggettivamente ingiustificato. Su tali presupposti, l'interrogazione del senatore Compagna è stata dal Presidente ritenuta ammissibile, annunciata e pubblicata nei Resoconti della seduta del 25 gennaio 2011. Il Governo, nella sua piena autonomia, ha espresso la propria volontà di rispondere alla stessa interrogazione nella seduta odierna, già precedentemente prevista dal calendario dei lavori per l'esame di strumenti di sindacato ispettivo. La Presidenza non poteva che prenderne atto. Con riferimento alla qualificazione di urgenza dell'interrogazione, la Presidenza, per prassi consolidata, non giudica sull'autoqualificazione dell'atto da parte del proponente. L'articolo 151 del Regolamento attribuisce piuttosto al Presidente la potestà di disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo ove non sia prevista un'apposita seduta dedicata allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dal comma 3 dell'articolo 148 del Regolamento. Tale norma consente al Governo di dichiarare all'Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato. In questo caso, tuttavia, la Presidenza ha solo preso atto dell'intenzione manifestata dal Governo di rispondere all'interrogazione in questione nella seduta di oggi che, come ho già ricordato, era già stata dedicata, secondo il calendario vigente, allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze. Allo stesso modo si è regolata la Presidenza per alcune interrogazioni urgenti presentate nel pomeriggio di ieri, anch'esse rivolte al Ministro degli affari, dopo averne acquisita la disponibilità.

affari esteri*. Signora Presidente, onorevoli senatori, è assolutamente essenziale che prima di rispondere nel merito alla prima delle quattro interrogazioni previste per la seduta odierna io svolga una precisazione sul metodo, avendo ascoltato, ovviamente, il dibattito sul Regolamento. Lo dico anzitutto alla presidente Finocchiaro: il Ministro degli affari esteri non si scomoda mai quando viene in Parlamento, fa semplicemente il suo dovere. Io stesso sono stato personalmente ascoltato dal Parlamento nelle scorse settimane, non una ma molte volte, su questioni urgenti,

Credo che un punto sia assolutamente chiaro: il Governo non può e non deve decidere se e dove essere ascoltato, in quale Camera, se in Commissione oppure in Aula. Oggi vengo chiamato in Aula su quattro interrogazioni e ritengo che sia mio dovere essere qui. Non assumerò mai

Come tutti ricorderanno, la scorsa estate è sorta un'accesa polemica sulla vicenda riguardante la proprietà di un appartamento situato a Montecarlo, già facente parte di un legato ad un partito politico italiano, Alleanza Nazionale, che si trovava nella disponibilità materiale di un cittadino italiano, Giancarlo Tulliani. Oggetto della polemica sono state anche l'origine e l'autenticità di un documento a firma del Ministro della giustizia di Santa Lucia, che attribuiva allo stesso signor Giancarlo Tulliani la titolarità di società *offshore* intestatarie dell'immobile. In detto documento, si sarebbe precisata e indicata l'esistenza di un'inchiesta disposta dalle autorità di Santa Lucia, nata dalla circostanza di dover accertare perché il prezzo di vendita di quell'appartamento fosse basso, in relazione al livello medio del prezzo di mercato di immobili collocati in Montecarlo. Vi fu una polemica una polemica che investì anche una presunta manipolazione del documento e quindi la sua autenticità; da alcuni organi di stampa, si era indicato anche un presunto ruolo di organi dello Stato in tali attività. Ecco la ragione per cui, a suo tempo, ritenni di chiedere, non ovviamente una rogatoria, ma un chiarimento puro e semplice alle autorità di Santa Lucia circa la genesi e l'autenticità del predetto documento, pubblicato da organi di informazione in Italia, e non solo in Italia, onde fugare dubbi, indiscrezioni, retroscena. Alcune settimane fa, ho ricevuto una risposta dal Primo Ministro di Santa Lucia, il quale, allegando il documento a suo tempo prodotto a lui stesso dal Ministro della giustizia, me ne ha certificato l'autenticità, e la veridicità dei dati in esso contenuti. Sia la lettera, sia il documento allegato sono stati da me inviati, per le valutazioni di competenza - e quindi non nell'indicazione di eventuali fattispecie di illecito, o di illecito penale alla procura della Repubblica di Roma, poiché mi risulta che vi sia ancora un fascicolo aperto sulla vicenda. Lasciando quindi agli organi giurisdizionali ogni valutazione di loro competenza, mi limito oggi a ribadire quanto vi ho appena detto. Il documento ovviamente non può essere messo ad integrale disposizione, e quindi sui particolari di questo documento

Signor Presidente, signor Ministro, nel prendere atto delle affermazioni del Governo, mi preme rilevare come la vicenda internazionale dipanatasi negli ultimi mesi tra il Principato monegasco e l'isola di Santa Lucia su cui era incentrato il mio atto di sindacato ispettivo ha acquisito nel corso di questi mesi un profilo istituzionale a mio giudizio improprio, che spero possa ora diradarsi grazie alla linearità degli argomenti di metodo fatta valere qualche minuto fa dall'onorevole Ministro. Instancabili protagonisti del cosiddetto giornalismo investigativo avevano ricamato e continuano a ricamare su questa vicenda con accanimento. Direi che c'è un tipo di giornalismo investigativo, che qualche volta mi viene da definire quello dei centrocampisti di Procura, cioè quel copia ed incolla che ha come fonte il terzo potere e, come dissi quando discutevamo un disegno di legge sulle intercettazioni, ha il suo eroe eponimo: parlo del giornalismo alla D'Avanzo. il giornalismo investigativo più liberale, più liberistico, più scollacciato, più spregiudicato - quello di Feltri - che ha iniziato ad animare fin dal luglio-agosto la vicenda, alimentandone per proprio conto profili di diceria, di insinuazione, di pettegolezzo. È poi comparso un terzo tipo di giornalismo investigativo, quello che vorrebbe avere un ruolo parastatuale. Vi è un agilissimo (non so se anche abilissimo) giornalista-editore che ha cercato di rivendicare per sé un ruolo parastatuale di indagatore su questa vicenda (mi riferisco alle vicende di ottobre). Da questo punto di vista ho ritenuto che un percorso istituzionale più nitido dovesse svolgersi, certamente in procura se ha detto bene il ministro Frattini - la procura lo riterrà. E lì i miei sentimenti non hanno nulla della mancanza di rispetto, di affetto, oltre ovviamente che per l'amico collega Pontone, per il Presidente della Camera, per il suo diritto alla trasparenza. Da questo punto di vista credo di dover prendere atto che proprio quest'appuntamento parlamentare, tanto contestato da alcuni colleghi, ha inteso riprodurre un clima più pacato, un clima di garanzie. Del resto, se posso concludere, colleghi, con una battuta sdrammatizzante, siamo quasi a metà, o a un po' più della metà, di questa legislatura. Francamente, non è mai stata l'Aula del Senato a investire o ad aggredire prerogative, ordini del giorno, calendari dell'altro ramo del Parlamento. E così, mi onoro - se poi ho sbagliato, ne porterò l'ignominia nella storia del Senato - di aver contribuito con questo atto di sindacato ispettivo (esprimendo

frequentemente sull'evoluzione della situazione nei Paesi del Nordafrica, in particolare del Maghreb. La scorsa settimana, come accennavo prima, ho avuto un lungo incontro con le Commissioni congiunte di Camera e Senato, mi ero riservato di tornare in Parlamento: quindi, l'occasione di oggi è utile, anche perché l'evoluzione della situazione in Egitto, in Tunisia, in Algeria e, recentemente, in Libano merita qualche riflessione, anzitutto informativa, e poi qualche proposta. In primo luogo, posso dare agli onorevoli senatori un aggiornamento di stamani, che arriva dalla nostra ambasciata Il Cairo. Alle ore 9 circa di questa mattina ci viene data notizia di una situazione sostanzialmente di calma apparente nelle aree dove ieri e l'altro ieri vi erano stati scontri, e questo sia al Cairo, sia nella zona di Suez. L'esito complessivo delle operazioni di polizia ha portato ad alcune centinaia di arresti. Vi sono purtroppo sei morti, di cui un agente di polizia. Di questi sei morti, tre sono a Suez, città che noi consideriamo con una situazione particolarmente calda, anche perché l'organizzazione dei Fratelli musulmani ha da oggi formalmente dichiarato di voler aderire all'organizzazione delle manifestazioni e delle proteste di piazza, particolarmente nella città di Suez. Una prospettiva nelle prossime ore è quella di un tentativo di avere nuove manifestazioni di piazza, particolarmente nelle zone centrali del Cairo, anche se le forze di polizia hanno vietato l'organizzazione di manifestazioni non formalmente autorizzate. Certamente, si immagina che la giornata di domani, giornata festiva, in particolare nelle ore che seguiranno la preghiera di fine mattinata, potrebbe essere una giornata particolarmente delicata. Ho ieri incontrato a Roma il ministro egiziano per lo sviluppo Rachid, in preparazione del vertice bilaterale Italia-Egitto che si svolgerà a metà di febbraio a Luxor. Il ministro Rachid ha descritto una condizione in cui il Governo egiziano intende non limitare la libertà di espressione e la libertà di informazione, né la libertà di associazione e manifestazione pacifica, cosa che ovviamente ha ricevuto da parte mia un incoraggiamento affinché sia consentito il normale svolgimento di un'informazione pubblica che, come voi sapete, in Egitto è garantita da 300 quotidiani. Vi è un problema serio alla base dei disordini, sia in Egitto sia in altre città del Maghreb e dell'Africa settentrionale. Sono le conseguenze, affrontate in ritardo e probabilmente non con provvedimenti organici, della crisi economica globale, che ha colpito soprattutto le fasce più povere, anche se in queste manifestazioni noi abbiamo visto nelle piazze, non solamente in Egitto ma anche in Tunisia, la presenza di persone appartenenti alle più diverse categorie della società e, quindi, anche professionisti, operai, lavoratori agricoli, e non soltanto disoccupati, come era nelle prime ore. Non pensiamo che, al di là di quanto sinora è accaduto, vi siano regie organizzate di formazioni dell'estremismo islamico più radicale; il fatto nuovo dell'adesione dei Fratelli musulmani d'Egitto alle manifestazioni introduce però un elemento di preoccupazione che fino a ieri, evidentemente, non c'era. Sono in programma delle manifestazioni, che seguiranno quelle dei giorni scorsi ad Alessandria e, come detto, anche a Suez. Non risulta in Egitto il coinvolgimento, né in ferimenti, né, peggio, in aggressioni di nostri connazionali. L'ambasciata d'Italia ha ovviamente invitato i connazionali alla massima cautela, attivando una rete di informazione tramite SMS sui cellulari di ciascuno degli italiani oggi presenti in quello Stato. Un luogo caldo delle manifestazioni di ieri è stata la zona vicina alla cancelleria consolare italiana, si trova vicino a piazza Tahir, una delle piazze ove sono avvenute manifestazioni. In alcuni momenti, effettivamente, la situazione è sfuggita al controllo delle forze di polizia, e alcuni lacrimogeni e sassi sono arrivati dentro il cortile del consolato. Per cautela oggi sono state sospese le attività della scuola italiana Leonardo da Vinci, che nel palazzo della cancelleria consolare. La situazione egiziana è in evoluzione,

Vi è stata una mobilitazione sostanzialmente unitaria dei manifestanti e dei dimostranti, che ha visto insieme persone di religioni diverse, appartenenti a diverse classi sociali, come detto, ivi compresi gli studenti universitari, e certamente questo impone - lo ha già imposto da parte dell'Unione europea, ma evidentemente lo impone anche da parte dell'Italia - un invito alla moderazione. Per quanto riguarda l'Egitto, confermiamo la profonda amicizia che lega il popolo italiano al popolo egiziano e riteniamo interesse prioritario dell'Italia e dell'Europa la stabilità di questo Paese. L'Egitto è un partner insostituibile dell'Europa e della comunità internazionale nel Mediterraneo, ed è anche un attore estremamente importante che, come voi sapete, svolge un ruolo di grande moderazione sia per la riconciliazione interpalestinese, sia per il processo di pace tra palestinesi e israeliani.

Diversa è la situazione in Tunisia, perché nata da motivazioni sostanzialmente differenti, anche se pure in quel Paese non si può parlare

vi è stato un malcontento crescente verso la classe dirigente tunisina, non solo verso il Governo, in particolare per le carenze nel Paese in materia di godimento delle libertà politiche e civili. Una delle ragioni che ha scatenato la protesta tunisina è il forte squilibrio territoriale esistente tra regioni arretrate del Sud-Ovest e dell'interno del Paese e la zona più ricca dell'area costiera della Tunisia.

ad un ulteriore forte rimpasto del Governo tunisino che dovrebbe riguardare alcuni dei Ministri i con portafogli più importanti dell'attuale Governo transitorio. L'obiettivo è accompagnare la crescita economica, che certamente vi è stata, con un'evoluzione parallela, in senso democratico, delle istituzioni e con un ricambio generazionale della classe dirigente. Questo è il punto che ha fatto mettere al centro della protesta tunisina il tema della corruzione e della difficoltà di collaborazione tra l'Esercito, che ha dimostrato lealtà all'assetto costituzionale, e una parte della Polizia e delle forze di sicurezza, che hanno invece svolto un ruolo talvolta di vere e proprie milizie già appartenenti alla guardia presidenziale. Certamente, anche la Tunisia ha una potenziale vulnerabilità, che ancora non si è manifestata, relativa all'interesse evidente di gruppi terroristici collegati ad Al-Qaeda Sahara (un'organizzazione che purtroppo esiste da tempo e che si dedica al traffico di armi, di droga, a sequestri di persona), che certamente nella vulnerabilità

Governo di cui dicevo, vi è una forte richiesta per la costituzione di un cosiddetto comitato dei saggi, che potrebbe reggere il Paese fino allo svolgimento delle libere elezioni. Il recente avvio di un'inchiesta internazionale con il mandato d'arresto nei confronti del presidente Ben Ali e di alcuni familiari ha aperto un ulteriore fronte nel quadro della lotta dell'attuale Governo transitorio contro la corruzione, questione che ovviamente noi pensiamo sia uno dei punti chiave dai quali partire per rilanciare la situazione politica interna ed istituzionale tunisina.

finora fuorilegge o comunque marginalizzati, dovranno essere messi in condizione di strutturarsi sul territorio per acquisire rappresentatività. Diversa la situazione in Algeria. Le manifestazioni popolari in Algeria si sono diffuse da Algeri in gran parte del Paese; il Governo algerino ha adottato alcune misure rapide, di tipo economico, sulla gestione e l'andamento dei prezzi di prodotti alimentari quali l'olio e lo zucchero, che avevano determinato le proteste.

con arresti di alcuni autori e promotori del movimento di protesta. La gran parte della popolazione ha condiviso

in occasione del 19° anniversario dell'entrata in vigore dello stato di emergenza. Sarà una manifestazione simbolica di questa data: quindi, dal 9 febbraio in poi vi è l'annuncio di una manifestazione.

l'attrazione fondamentalista, tanto che i leader storici del movimento fondamentalista hanno tentato senza successo - io dico fortunatamente - di mobilitare i rivoltosi. Ecco quindi che in tutti questi Paesi - per passare all'analisi e alla proposta - vi è stato quello che il Segretario generale della Lega araba ha opportunamente definito uno «*shock* sociale», la necessità di aprire alla società civile e di comprendere il bisogno di modernizzazione e di democratizzazione, senza commettere però l'errore, che noi europei non dobbiamo e non possiamo permetterci, di indicare dall'Europa quale sia la strada giusta da imboccare, quale sia la ricetta ed il modello. Questo sarebbe ad avviso della stessa Lega araba - e io dico: giustamente - un tentativo di stampo quasi post-coloniale di indirizzare e di proporre soluzioni preconfezionate altrove. Sarebbe sbagliato, anche perché, da Paese a Paese, la storia, la cultura e le tradizioni sono diverse. Vi è allora la necessità di partire anzitutto da un'azione europea, di cui ho avuto occasione di parlare già

del Sud del Mediterraneo, cui l'Italia guarda con attenzione prioritaria. Una prima idea che ho ventilato, e che spero si tradurrà presto in realtà, la costituzione di una delegazione europea di alto livello, che possa inviare una missione europea in ciascuno di questi Paesi, per prendere contatto ai più alti livelli, a partire dalle autorità tunisine, con la società civile, con i sindacati, con i partiti di opposizione, ovviamente per raccogliere informazioni, e non certo per dare prescrizioni. Credo che

l'Europa possa e debba proporre un'assistenza - se richiesta, evidentemente: non la andremo certamente ad imporre - ed un *team* di monitoraggio per accompagnare lo svolgimento delle elezioni. La terza iniziativa che credo l'Europa debba avviare, in consultazione con il Governo tunisino, è l'adozione di misure restrittive europee nei confronti di individui appartenenti al passato regime (si è parlato del congelamento degli assetti patrimoniali). Non ritengo si possa trattare di iniziative sporadiche di questo o di quel Paese dell'Europa, ma di un'iniziativa europea. Il Governo tunisino ha adottato un'iniziativa per istituire una commissione sui fenomeni di corruzione e sulle modalità delle violenze delle scorse settimane: se richiesta, credo che l'Europa debba fornire volentieri la propria assistenza anche di tipo tecnico. Evidentemente, vi è un altro strumento che possiamo utilizzare: com'è noto, la Tunisia, in particolare,

settentrionale mediterranea, proprio perché solo l'avvicinamento alla dimensione europea può essere un antidoto preventivo all'ulteriore manifestarsi di instabilità, di violenze e di contrasti. Credo che al riguardo l'Europa possa giocare sia sull'assistenza economico-finanziaria sia sull'assistenza politica, chiedendo evidentemente che nel quadro generale siano considerati i diritti umani e le libertà civili.

cinque Paesi della riva Sud mediterranea e cinque Paesi europei della riva Nord: quest'anno l'Italia ha la presidenza del relativo esercizio. Metteremo, dunque, tale esercizio al servizio di un'analisi mediterranea comune con questi Paesi (i 5+5), ma anche nella formula più allargata dell'Euromed. Riteniamo, quindi, che nelle prossime settimane l'Europa debba e possa, con il convinto sostegno dell'Italia, non solo seguire le vicende, ma anche intervenire con forza come Europa per evitare

più sviluppo nei Paesi di origine e, ancora una volta, che l'Europa si faccia carico di progetti economico-finanziari per evitare condizioni di povertà e talvolta di disperazione, ma al tempo stesso - è una cosa cui personalmente tengo molto - per favorire la mobilità, cioè la circolazione di giovani nel Mediterraneo. ho proposto una sorta di progetto Erasmus euromediterraneo, per consentire ai giovani delle università dei Paesi mediterranei del Sud maggiori possibilità di accesso alle opportunità di formazione nei Paesi mediterranei del Nord e dell'Europa, al fine di creare un altro fattore positivo per le giovani classi dirigenti di quei Paesi.

infatti dovuto approfittare della vicenda della casa di Montecarlo per poter parlare di una questione che riguarda il nostro Paese, i suoi interessi strategici, la sicurezza ed il futuro dei nostri connazionali che vivono in Algeria, in Egitto, in Tunisia ed in Libano - dove peraltro abbiamo una missione

Devo dirle che le priorità di questo Governo non sono quelle che dovrebbero essere, perché la priorità è di rendere al Parlamento un'informativa su questa materia e non quella di rendersi strumento più o meno inconsapevole di lotta politica. Vorrei qui aprire una parentesi: forse lei non si è reso conto di ciò che ha fatto con l'atto di trasmissione di queste carte alla procura di Roma. Se infatti queste carte non hanno alcun rilievo per l'indagine penale,

dal diritto internazionale e dalla legge sulle rogatorie (che è stata modificata peraltro nella legislatura 2001-2006 proprio per consentire la genuinità dell'acquisizione di determinati atti probatori provenienti dall'estero

si sia resa strumento di una vicenda indecente, che non fa onore alla politica italiana, a questo Governo e a questa maggioranza, che sono ormai alla canna del gas. Per quanto riguarda l'informativa, noi prendiamo atto Grazie

Sarà una strana coincidenza che in Libano, come anche in Tunisia, in Egitto e in Algeria, la gente manifesti, si mobiliti, scenda in piazza per protestare contro Governi che hanno violato e violano sistematicamente diritti umani

e l'integralismo diventi una miscela esplosiva, che ci fa trovare Paese confinante con altri Stati che possono cambiare in peggio la loro *leadership* politica ed istituzionale. ci fa preoccupare ulteriormente: infatti, se in Tunisia si è scelta la strada di perseguire penalmente il presidente Ben Ali e la sua famiglia, e lo si è fatto con un mandato di cattura internazionale, significa che la situazione di scontro sociale in quel Paese è così forte che neanche le soluzioni politiche, più o meno moderate, che sono state trovate in queste settimane riescono a calmare le popolazioni. stessa situazione rischia di verificarsi in Egitto. Capisco quindi la necessità di continuare l'interlocuzione con il Governo egiziano fin quando c'è, e ci auguriamo che ci sia, perché, se un cambio ci deve essere nella *leadership* di questi Governi, esso avvenga assecondando le *leadership* moderate di quei Paesi, e avvenga con un'iniziativa forte, intanto dell'Italia, delegarla solo all'Unione europea significherebbe allungare i tempi. Infatti, il primo Paese di frontiera siamo noi, che abbiamo poi il problema dell'immigrazione da questi Paesi, dalla Tunisia, come dall'Egitto: immigrazione alla quale non siamo preparati e rispetto alla quale il Governo non dice nulla e non ci dà alcuna ipotesi di soluzione, ma che avverrà, come sta in parte avvenendo. Inoltre, noi abbiamo fortissimi interessi economici concentrati in quei Paesi, che devono indurci ad assumere iniziative, certamente nel quadro dell'Unione europea: ma il conto per primi lo paghiamo noi, e quindi abbiamo bisogno che il nostro Paese sia in prima fila rispetto alle questioni riguardanti il Mediterraneo. Da questo punto di vista, prendiamo atto della sua informativa, ma ritengo che su tali questioni dovremmo ritornare, magari in Commissione, per seguire e monitorare settimanalmente quanto succede, proprio per l'urgenza di avere una posizione chiara da parte del nostro Paese.

senza fattori nazionali che implicano problematiche internazionali, forse l'Italia potrebbe riprendere il ruolo che svolgeva una volta nel Mediterraneo Grazie

anche pensare a quello che può essere il bacino di un vero problema nel Mediterraneo, un vero germe che sta per nascere. Se pensa al fattore di tutti questi Paesi che stanno iniziando a ribellarsi, essi hanno in sé, e lei lo sa, signor Ministro,

attraverso gli Stati Uniti (e questa volta sono obbligata a dirlo, nonostante io sia molto amica dei colleghi americani), abbiamo promosso, o comunque accettato la divisione del più grande Stato africano, il Sudan. Io ritengo che questo sia stato un grandissimo errore

*(IdV)*. Signor Presidente, signor Ministro, ciò che ha dichiarato oggi sui problemi del Nordafrica, sulla Tunisia, sull'Algeria è quanto è stato riportato in questi giorni dai quotidiani.

Ha fatto un «copia e incolla» che non serve a nulla: solo a giustificare la sua presenza per rispondere e dare un segnale intimidatorio a qualche ex compagno di avventura. questo mi dispiace, visto che lei dovrebbe pensare più alla politica estera che non a diatribe interne. a questi Paesi del Nordafrica, come ha detto la collega Contini, dopo la calma solo apparente di questi giorni, ieri i tunisini sono tornati a manifestare a Sfax anche contro il nuovo Primo Ministro, accusato di essere stato sempre e comunque alleato di Ben Ali. Ben Ali. Ieri, in conferenza stampa, sono state annunciate le cifre di un mese di «rivolta del gelsomino»: 700 arresti, 74 detenuti in carcere e ben 11.000 evasi. Il tutto mentre, su richiesta del Governo *ad interim*, veniva diramato dall'Interpol un mandato di arresto internazionale nei confronti di Ben Ali, la moglie, il cognato e altri otto appartenenti al *clan* del deposto Presidente. L'accusa è l'indebita acquisizione di beni mobili e immobili, oltre che il trasferimento illecito di valuta all'estero. È innegabile che, alla base degli scontri, vi siano anche movimenti politici e geopolitici, ma il moto propulsivo per la rivolta è stato socio-economico: una popolazione in grave stato di povertà, nonostante gli enormi introiti petroliferi dello Stato; una disparità sociale elevatissima e la mancanza di servizi pubblici diffusi. Anche queste caratteristiche sono presenti con forza nei restanti Paesi del Nordafrica, quali Marocco, Algeria, Libia ed Egitto. Pertanto, non possiamo escludere un effetto domino. Il caso Egitto, colleghi, in tutta la sua pericolosità, è sotto gli occhi di tutti. Ancora oggi sono forti gli scontri, centinaia gli arresti. Nella sola giornata

al figlio vero di Mubarak, e non voglio scendere a simpatiche illazioni (ma lei ha capito a che cosa mi riferisco). Da lei, signor Ministro, avrei voluto sapere se abbiamo avviato relazioni bilaterali e se l'Esecutivo tenga rapporti non soltanto con i Governi ma anche con tutte le associazioni: quelle associazioni economiche e politiche che si propongono come alternative dei Governi in carica, situate sia nei Paesi del Maghreb che in Italia. Italia. Signor Ministro, avrei voluto che nel suo intervento avessero trovato spazio dei chiarimenti sulle relazioni privilegiate che Berlusconi intrattiene con il dittatore Gheddafi, sulla sudditanza economica e la dipendenza dal punto di vista dell'immigrazione. E qui si possono mettere dei limiti alla nostra libertà di azione, preoccupazione è ampiamente giustificata leggendo sui giornali e in base alle iniziative che voi supinamente avete subito da questo dittatore. Mi riferisco ai limiti alla nostra libertà d'azione e di discrezionalità politica, visto che il Rais ha sostenuto il 15 gennaio: «Mi dispiace per Ben Ali».

Purtroppo ieri il suo Dicastero - sempre da quanto si apprende dalla stampa - sarebbe stato più impegnato a ricevere le carte che giungevano da un altro piccolo Stato, dei Caraibi, retto da amici personali, quanto non soci di affari del Presidente del Consiglio. Presenterò poi un'altra interrogazione parlamentare, quando sarà - vedremo se ci sarà la stessa celerità odierna - su che cosa ha comportato l'acquisto delle case in Antigua, su quali sono le società *offshore* dietro a quelle vendite, chi ha acquistato, quali società sono intervenute, e chiederò - forse delegheranno sempre lei anche di sapere quanto sono costate le case alle "olgettine", quanto pagavano gli affittuari di cui in questi giorni leggiamo sui giornali. Vogliamo leggere i contratti, le dichiarazioni che ogni affittuario, come prevede la legge Moro, ha dovuto consegnare ai carabinieri. Credo che anche su questo delegheranno lei per la risposta.

l'informativa che questa mattina ha svolto il signor ministro Frattini, che ringraziamo per la sua puntuale e precisa illustrazione di una situazione di fatto e per aver delineato le strategie di intervento che il suo Ministero vuole attuare in queste circostanze, e le interrogazioni presentate dai colleghi senatori ci consentono di di svolgere nostre considerazioni, seppure brevi, su quanto sta succedendo in tutti i Paesi del Nordafrica, e non solo (cito ad esempio l'Albania, a noi vicina). Noi siamo molto preoccupati per tutto

Alla fine, signor Ministro e illustri colleghi, quelli che ci rimettono sono sempre i poveri diavoli. Abbiamo ricordato proprio in quest'Aula qualche settimana fa la strage dei cristiani avvenuta in Egitto.

Insomma, è iniziato un proliferare di focolai di guerra che potrebbero scatenare reazioni a catena e coinvolgere anche altri Paesi. La Lega Nord chiede semplicemente al signor Ministro e al Governo il massimo impegno, nella piena consapevolezza che ciò sta già avvenendo, per cercare di garantire con tutte le armi della diplomazia che si hanno a disposizione la stabilità e la sicurezza di questi Paesi. Le cosiddette guerre civili sono sempre le più sanguinose, anche perché in alcuni Paesi cosiddetti poveri l'interesse mediatico lascia molto a desiderare, forse perché non ci sono interessi economici e commerciali. L'instabilità di questi Paesi favorisce la disperazione, la fuga, l'emigrazione clandestina, sfruttata poi, come al solito, dalla criminalità organizzata o da quelle frange religiose estremiste di terroristi islamici che condizionano negativamente la vita di altri Paesi, compreso il nostro. In conclusione, signor Ministro,

sul lavoro delle nostre ambasciate e dei nostri consolati affinché sia sempre compiuto nell'interesse dei nostri connazionali residenti in quei Paesi

Signor Presidente, signor Ministro, quando ieri abbiamo appreso dalle agenzie di stampa che sarebbe venuto qui in Senato per rispondere ad una interrogazione urgente del senatore Compagna presentata poche ore prima, come Gruppo abbiamo riflettuto sulla dignità e il decoro delle istituzioni, che in un momento come questo non potevano consentire che il Ministro degli affari esteri venisse in Senato per discutere soltanto di una questione riguardante sostanzialmente la vita privata del Presidente della Camera, senza fare il punto il punto su argomenti di ben altro rilievo, quali le tensioni, che lei ha descritto con parole molto accurate, in tutta la riva Sud del Mediterraneo e sugli impegni che l'Italia intende assolvere rispetto a tale questione, essendo il nostro il Paese che più degli altri si trova al centro e nel cuore

un allargamento dell'ordine del giorno, e le siamo grati per aver voluto tenere questa relazione. Una relazione che giudichiamo ragionevole ed esauriente dal punto di vista descrittivo. Tuttavia, signor Ministro, vorremmo che il nostro Governo facesse qualcosa di più, Governo facesse qualcosa di più, innanzitutto sotto il profilo dell'analisi. Lei ha descritto molto bene tutti gli aspetti delle varie crisi in corso, ma c'è un punto che accomuna

che è anche demografica, in quei Paesi - che si va saldando con una questione democratica e che rischia di saldarsi con quella religiosa. Se questi tre elementi dovessero mettersi insieme, è evidente che assisteremmo ad un vero e proprio incendio nella riva Sud del Mediterraneo e dovremmo aspettarci di convivere con regimi che potrebbero essere aggressivi e pericolosi. Lei ha giustamente detto che la stabilità è un valore, come è un impegno necessario la lotta contro il fondamentalismo. Tuttavia, questa situazione ci dice che oggi non è possibile immaginare nessuna stabilità senza un quadro, una cornice di evoluzione democratica di quei Paesi. Lei ha giustamente detto, e noi lo condividiamo, che dobbiamo mettere al bando qualunque tentazione di tipo neocoloniale, che

dei Paesi arabi e islamici. Non è questo il nostro intento. Il punto fondamentale è che i popoli di quei Paesi devono sentire l'Europa e l'Italia vicine,

(non a caso lei è a capo della nostra diplomazia), deve esserci anche la nettezza, il coraggio, la *moral suasion* nei confronti dei regimi di quei Paesi, perché si mettano su una strada di progressiva evoluzione democratica.

economico - con quei popoli, nella ricerca di una loro via per la libertà. Potremmo altrimenti correre il rischio di trovarci di fronte a situazioni difficili, come quella che oggi dobbiamo fronteggiare in Tunisia, dove

troppo e troppo a lungo (fino agli ultimi giorni, dando anche prova di avere sensori imperfetti della situazione sul campo) i sostenitori di un regime che oggi è

decise liberamente dal popolo, con libere elezioni tra sei mesi. Questo dovrebbe esserci da insegnamento anche rispetto agli altri Paesi e alle altre situazioni della riva Sud del Mediterraneo, che resta per noi un interlocutore assolutamente strategico ed è una delle aree nevralgiche per la pace nel mondo.

sempre puntuale non solo in Aula ma anche in Commissione per darci il sentimento del Governo su tutto quello che succede a livello internazionale, e non per dirci soltanto dei fatti che si leggono sulla stampa, come è stato detto poco fa. Infatti, quello che ci ha detto il Ministro è anche la descrizione di un impegno del Governo italiano rinnovato e una filosofia di impegno in queste aree che, a partire dalla prossima riunione a Napoli di cui ci ha dato notizia, potrebbe sottolineare un rinnovato ruolo del nostro Paese in un'area che

come è stato rilevato da qualcuno che ha fatto un commento più politologico che politico di questo avvenimento, ma che ha secondo me centrato l'argomento, con la Tunisia è finito il mito della piazza araba eternamente in subbuglio per il suo atteggiamento antioccidentale. Io credo che la rivoluzione tunisina - chiamiamola così per capirci meglio - abbia spazzato via una delle immagini meno confortevoli che hanno distinto il Medio Oriente da più di cinquant'anni, cioè quella di una piazza araba eccitata dall'antisemitismo e dall'odio per gli Stati Uniti in particolare, ma incapace di avere un avere un vero senso rinnovatore al proprio interno, nei confronti dei propri governanti. Noi abbiamo visto molte volte dei movimenti non certamente tranquilli in Tunisia per l'indigenza, la scarsità di mezzi di sussistenza, per le partite di calcio, per tutto quello che aveva e ha sempre avuto una inconcludenza, una scarsa presa dal punto di vista del profilo politico di questi movimenti. Adesso credo che sia cambiata la filosofia e il modo di agire. Quanto Quanto succede in Tunisia credo abbia la forza di un cambiamento anche all'interno di quel Paese e soprattutto la possibilità di avere un effetto domino - e questo non è positivo

questo è particolarmente preoccupante, perché la stabilità dell'Egitto è strategica per la questione palestinese, per l'egemonia iraniana e anche per tutta l'area mediorientale. Io credo che la stabilità dell'Egitto sia sempre stata uno dei punti cui il nostro Governo ha guardato con particolare attenzione, non solo perché è un Paese *partner* dell'Italia ma anche perché consente, o ha consentito in questi ultimi tempi una certa tolleranza per quanto riguarda lo stato d'animo della propria popolazione, e soprattutto - questo è un tema che mi è molto caro, e apprezzo particolarmente quello che ci ha detto il Ministro - per l'Europa e il ruolo e l'azione che l'Europa deve svolgere. ho sempre insistito, da qualche anno a questa parte, sul fatto che l'Europa deve recuperare un ruolo politico nel contesto internazionale. Non può permettersi il lusso di un'azione *a* *posteriori*: deve prendere l'iniziativa e svolgere un ruolo di negoziato e di aiuto, ma anche di *leadership* politica. Ci ha detto, signor Ministro, delle prossime tappe che centrano sull'Europa l'attenzione del nostro Governo, ma anche di tanti altri Paesi che dall'Unione europea si aspettano un impulso, non soltanto in termini di aiuti economici, ma anche di civiltà politica, che abbiamo il dovere di dare a questi Paesi:

Signor Presidente, signor Ministro, io e altri firmatari abbiamo chiesto circa a metà novembre perché

a differenza del settore privato, un rapporto che, nonostante la rottura delle relazioni sindacali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è migliore e più proficuo.

- ma anche se ci sono stati interventi esterni, e vogliamo soprattutto sapere quando si faranno le prossime elezioni. Questo, perché nell'accordo del pubblico impiego quella legge segna per le organizzazioni sindacali un punto d'approdo molto importante, anche per un accordo sulla rappresentanza che i fatti ultimi della FIAT rendono ancora ancora più importante. Potrebbe avere un effetto benefico rispetto a un processo di unità. Vogliamo saperlo anche perché ci sono cose che non ci convincono. Sarò molto franco con lei. Parto da una notizia di giornale che non riguarda il pubblico impiego: quando il segretario dell'UGL dice che ha più iscritti della UIL di Angeletti

come era nel 1992 prima che l'allora sottosegretario Sacconi iniziasse una procedura che poi fu conclusa da Bassanini e D'Antona, abbia gli stessi poteri e le stesse risorse economiche

meglio di me che c'è, questa idea di non avere nessun controllo, in un momento in cui i sindacati hanno una funzione importante, sia sul terreno della sussidiarietà, con la bilateralità, sia anche in una

e quanto fu faticoso con il Governo Amato, e poi per i Governi successivi, di Ciampi, Dini e Prodi, diradare questo bosco non corretto.

e anche questo apre la strada a quella preoccupazione che le dicevo: torniamo al passato, dove ognuno si arrangia per i fatti suoi, anche aprendo un possibile contenzioso di carattere economico, perché se a seguito di quella rappresentatività i sindacati più rappresentativi perdono risorse non è che taceranno. Io da lei non solo voglio sapere perché è accaduto, ma soprattutto cosa fa il Governo per andare rapidamente al ripristino di questa legge e di questo luogo democratico che sono le RSU e al ripristino delle regole, che peraltro, dal punto di vista contrattuale sono state applicate ma che, in un luogo dove ci sono oltre 16.000 punti di

Nel dare attuazione a tale previsione, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha disposto che siano definiti sino ad un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondano non più di quattro separate aree della dirigenza. È evidente la novità che tale previsione comporta rispetto al previgente sistema contrattuale, anche sotto il profilo dei soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione nazionale. In relazione a quest'ultimo aspetto, tuttavia, si sottolinea che le specifiche regole vigenti per il pubblico impiego in materia di rappresentatività sindacale non sono state ricomprese tra quelle oggetto di riordino della suindicata delega, di cui alla legge n. 15 del 2009. In proposito, com'è noto, la rappresentatività sindacale del pubblico impiego, disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede come soglia per la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale la percentuale non inferiore al 5 per cento nel comparto o nell'area, considerata come media tra il dato associativo e quello elettorale, cioè Il dato, associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato; quello elettorale, invece, è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, rispetto al totale dei voti espresso nell'ambito considerato. L'applicazione di tale disciplina alle nuove fasi contrattuali implica alcune conseguenze sostanziali, con particolare riferimento alla necessità della corretta verifica dei requisiti che le organizzazioni sindacali devono possedere per partecipare alla contrattazione collettiva, requisiti che per il pubblico impiego - a differenza del settore privato - sono condizioni necessarie ed imprescindibili. Proprio in ragione di tale specificità, l'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dettato norme transitorie sulle procedure per l'individuazione della partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative prevedendo, in particolare che: «In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree e le aree di contrattazione (...), l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative (...). Sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010». La predetta norma, quindi, è volta a prorogare le elezioni delle RSU al fine di consentire il rinnovo degli organismi di rappresentanza dopo l'accordo di composizione dei nuovi comparti. Per lo svolgimento delle successive elezioni, infatti, contestualmente alla proroga, devono ricorrere le due seguenti condizioni, strettamente correlate tra loro: del nuovo accordo sui comparti e aree di contrattazione; dall'altro, il rinnovo degli organismi di rappresentanza, «con riferimento ai nuovi comparti». Il termine temporale in cui procedere a tale rinnovo è individuato nel decorso 30 novembre 2010. Quanto al primo aspetto, si sottolinea che negli incontri tenutisi presso l'ARAN (l'Agenzia negoziale terza operante per il pubblico impiego) tutte le confederazioni sindacali presenti al confronto hanno evidenziato la necessità di definire, prima delle elezioni delle RSU, il nuovo accordo quadro sulla composizione dei nuovi comparti di contrattazione. Per quanto riguarda invece l'aspetto relativo al termine del 30 novembre 2010, le parti presenti al tavolo di confronto hanno espresso valutazioni differenti circa la perentorietà o meno del termine. Successivamente, dal mese di settembre 2010 ad oggi, sono stati convocati circa sette incontri presso l'ARAN al fine di definire la composizione dei nuovi comparti di contrattazione. La trattativa per la definizione dei nuovi comparti, tuttavia, è ancora in corso e non ha dato, finora, alcun esito. dato, finora, alcun esito. Relativamente all'interpretazione da dare al termine del 30 novembre 2010, si rileva che la proroga, contenuta nel citato articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, è finalizzata a consentire alle parti, in via transitoria ed in attesa della definizione di nuovi comparti, di mantenere una stretta correlazione tra composizione dei comparti e RSU. Ciò in quanto i risultati delle elezioni delle RSU non possono che essere collegati

sostanzialmente, cambierebbe la geografia della rappresentatività. Tale condizione assume pertanto un ruolo sostanziale, prevalente e prioritario rispetto allo stesso termine del 30 novembre 2010. Peraltro, successivamente il decreto-legge 30 dicembre 1994, n. 194, ha previsto che «ai fini della partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro

2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009». Conseguentemente - mi scuso per la complessità della trattazione, però era doverosa - la naturale scadenza del mandato degli organismi di rappresentanza in esame viene prorogata sino all'elezione dei nuovi rappresentanti delle RSU, anche ove essa avvenga oltre il termine del 30 novembre 2010. Quanto illustrato, in particolare per ciò che riguarda la proroga degli organismi di rappresentanza, non ha inteso, né intende determinare alcuna lesione del sistema contrattuale vigente. L'impianto normativo che ne emerge, così come le procedure negoziali sin qui promosse e percorse, viceversa, sono stati e sono tuttora finalizzati proprio a garantire, sulla base dei nuovi assetti di comparto derivanti dalla legittima autonomia negoziale, la più trasparente ed efficace procedura di rinnovo degli organismi di rappresentanza nel settore pubblico.

per questa fase transitoria il *mix* tra elezione e rappresentanza, e quindi vigilerà affinché non avvengano fatti che vanno contro questo *mix*, cioè azioni unilaterali dei soli iscritti,

Questo non può essere. Lei ha delle responsabilità: se ad un certo punto l'accordo non si fa, lei, che è così decisionista quando vuole, dovrà pur decidere in qualche modo - assieme, ovviamente, alle Regioni e ai Comuni, nell'ambito dei poteri che essi hanno

non va bene per quella legge che rappresenta un punto avanzatissimo dell'idea di rappresentanza, del *mix* di diverse culture sindacali, né va bene perché in questo modo non aiuteremmo i sindacati nel loro insieme a trovare una soluzione che riguarda

Avverte che i senatori Mariapia Garavaglia, Pedica e Spadoni Urbani hanno comunicato alla Presidenza di voler trasformare le interrogazioni all'ordine del giorno, di cui sono primi firmatari, in interrogazioni a risposta scritta.

Oggi è il Giorno della Memoria e ritengo che, se non vi fosse stato l'intervento del senatore Villari, che in effetti ha ristabilito un minimo di memoria storica sull'avvio di questa legislatura, si sarebbero ascoltate molte dichiarazioni da chi è complice di una totale mancanza di rispetto delle regole. La vicenda della Presidenza della Commissione di vigilanza Rai è sicuramente una ferita alla legalità costituzionale. Credo abbia fatto bene il senatore Villari a ricordarlo, sia pure brevemente. La memoria che oggi abbiamo voluto celebrare in quest'Aula purtroppo non appartiene al passato: esistono ancora persecuzioni, non più in virtù di un'appartenenza etnica, ma sempre più spesso in virtù di un'appartenenza religiosa e anche di un'identità di genere od orientamento sessuale. Ieri, alle ore 13, in Uganda, è stato trovato morto un iscritto all'associazione radicale «Certi diritti», un militante dei diritti *gay* che si chiamava David Kato, che nel novembre scorso avevamo invitato a Roma per presentare il libro sulla sua storia: la storia - appunto - di chi si batte in un Paese dove, purtroppo (non si tratta dell'unico caso nell'Africa sub-sahariana), l'omosessualità è considerata di per sé un reato, punibile con la reclusione David Kato, assieme ad altre 100 persone in Uganda, era stato incluso in un articolo della rivista locale «Rolling Stone», che metteva alla berlina per presunta omosessualità persone che avevano anche responsabilità all'interno della società ugandese.

il nostro Paese, assieme ad altri europei, è molto attento agli sviluppi in quello Stato. Spero che domani ai funerali vi sia una rappresentanza della nostra diplomazia in Uganda e che l'Italia partecipi in maniera attiva affinché le indagini possano portare alla luce i responsabili. Concludo suggerendo la visione di un video sul sito «Current TV», dove vi è - ahinoi - un'ulteriore strumentalizzazione della religione: predicatori evangelici che dicono «Dio odia i *gay*» ed una serie di manifestazioni di persecuzione quotidiana nei confronti di queste persone. Ricordiamoci che la memoria ci deve far continuare a denunciare le stragi del passato;

sollecitando la risposta alle numerose interrogazioni ed interpellanze che giacciono inevase da anni e che forse non saranno mai evase, nonostante non mi stanchi di sollecitare risposta quasi ad ogni fine seduta. Lungi da me alcuna polemica sulle case all'estero del cognato della terza carica dello Stato, ma vista la solerzia del Governo e del ministro Frattini, che torna in Senato dopo due anni per rispondere *ad horas* ad alcune interrogazioni, mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo su centinaia di atti di sindacato ispettivo

Chiedevo al Governo notizie sulla Flat Point Development, con sede legale ad Antigua, un Paese *offshore*, e una sede secondaria a Torino in galleria San Federico 54, di cui non si conosce il proprietario, così come non si conosce la motivazione dei 25 milioni di euro giunti in tre anni sul conto corrente della Flat Point, acceso presso la filiale milanese di Banca Arner, e subito trasferiti in Svizzera. La sede di Torino sarebbe il quartier generale italiano per raccogliere i clienti, anche se chiamando ad Antigua rimandano ad un sito Internet. La Banca Arner, tra l'altro, non è una banca qualsiasi, perché tra i suoi soci annovera, oltre a Nicola Bravetti, Paolo Del Bue, con il 34,8 per cento In tre anni, signor Presidente - e mi scuso se abuso sempre della sua pazienza alla fine della seduta, ma questo mi dà ancora più ragione, perché non ci sono senatori di serie A e di serie B in quel rapporto fiduciario sono passati 25 milioni di euro, soldi che venivano bonificati da banche italiane sul conto della Arner di Milano e poi quasi contemporaneamente trasferiti a Lugano. Grazie alla triangolazione con la sede milanese della Arner, si riusciva a evitare la normativa antiriciclaggio; così nel 2005 sono passati 1,8 milioni di euro sui conti della Flat Point, altri 343.000 nel 2006 e ben 13,1 milioni nel 2007. ben 13,1 milioni nel 2007. Questo flusso di denaro si è interrotto solo a giugno, quando nel registro degli indagati è finito lo stesso Marcheselli per favoreggiamento al riciclaggio. Da un'ispezione della Banca d'Italia sarebbe emersa l'impossibilità di accertare i beneficiari economici di alcune società che hanno il conto alla Arner Italia. Italia. Signor Presidente, se i senatori non sono ripartiti fra quelli di serie A, ai quali vengono date risposte immediate, e quelli di serie B, ai quali non vengono date affatto, sollecito il Governo a rispondere almeno a questa interrogazione vecchia di 13 mesi (senza pretendere di avere risposta immediata: